verso la società di cartolarizzazione dei crediti della previdenza sociale. Francamente non capisco l'ostilità quasi preconcetta nei riguardi di questo emendamento che, oltre tutto, non costa neanche un euro al Governo, anzi consentirebbe alla previdenza sociale di rientrare di alcuni crediti, perché gli agricoltori delle zone svantaggiate - non soltanto quelli del Meridione d'Italia, ma di tutte le zone svantaggiate chiedono semplicemente di mettersi in regola, con i tempi e i modi dovuti e secondo modalità che peraltro sono state già seguite da altri agricoltori,

tantissimi agricoltori, tante aziende, ma soprattutto tante famiglie.

oltre ad incidere sull'intero territorio nazionale, opera con riguardo ai quadri del Mezzogiorno, un adeguato finanziamento. Per far ciò, la proposta, condivisa dal collega Milana e che trova me come primo firmatario,

per dar vita ad una serie di attività formative che il Formez - che recentemente è stato, ad opera del ministro Brunetta, sdoppiato con l'istituzione di un segmento che più decisamente e precisamente si riferisce alla formazione, e che perciò

è stato un taglio consistente su questa parte, che è invece importante. Sappiamo che la salute dell'uomo è strettamente legata anche alla salute animale. in questi ultimi anni, abbiamo assistito sempre di più ad un aumento del randagismo, all'inselvatichimento di questi animali che non vengono più controllati sul territorio. Tagliare queste spese, secondo me, è un elemento di enorme gravità perché impedisce di affrontare tali questioni,

Il sostegno dell'editoria, come del resto anche all'emittenza privata, è un argomento molto sentito da tutte le forze di maggioranza e di opposizione, non solo perché gli stanziamenti in questi settori in questi settori sono indispensabili per assicurare il pluralismo dell'informazione, ma anche perché garantiscono un gran numero di posti di lavoro e sono anche uno strumento fondamentale di

una tremenda tromba d'aria, quasi un tornado, ha distrutto una grossa porzione della frazione di Vallà. Sono passati circa sei mesi ed il Governo

senatore Marcucci

a novembre in Italia nessun teatro - grande, medio o piccolo - conosce l'entità dei finanziamenti che avrà a disposizione. La stessa incertezza pesa sul complesso del mondo dello spettacolo, sul cinema, sulla musica, così come sul settore dei beni culturali, rischiando di compromettere, ad esempio, la fondamentale attività delle soprintendenze su tutto il territorio nazionale. A giudicare da quanto è stato fatto fino ad oggi, si può dire che questo Governo voglia abdicare a quella che è una funzione stabilita dalla nostra Costituzione e dalle leggi, vale a dire la tutela pubblica dei beni culturali.

la maggior parte delle riduzioni di spesa previste per il triennio 2009-2011 grava, infatti, sulla voce «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», vera e propria ragione sociale del Ministero.

Alla fine di questo percorso, praticamente resteranno sul bilancio del Collegio Romano solo gli stipendi del personale, del resto in via di dismissione, si considera che l'età media dei funzionari è intorno ai 55 anni e che le pochissime nuove assunzioni non coprono neanche il 10 per cento Questo è il cuore del problema che il Governo ha determinato e che il ministro Bondi sembra non contrastare. Purtroppo anche il parziale reintegro del FUS, dopo un anno di proteste *bipartisan*,in questo contesto sembra davvero poca cosa, perché ad una costante politica degli annunci, praticata con frequenza dal Ministro, non sono mai seguiti i fatti. Così, come Partito Democratico continuiamo a richiedere una profonda revisione dei tagli miopi che colpiscono la cultura, ma che vanno a limitare fortemente le potenzialità di sviluppo del nostro Paese. Chiediamo leggi di riforma vere, ad esempio per le fondazioni lirico-sinfoniche, la cui gravissima situazione di agonia viene praticamente ignorata. Voglio concludere citando le parole usate dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel corso della manifestazione che ho richiamato all'inizio del mio intervento: «Quando si parla di tagli, le cifre non dicono tutto e non tutte le voci di spesa sono uguali; bisogna confrontarsi nel merito delle conseguenze che può avere una decisione restrittiva, in particolare per settori come quello della cultura». È esattamente il confronto che chiediamo insistentemente al Governo, perché rifletta su una scelta che rischia di essere suicida per tutto il Paese, a dispetto delle chiacchiere.

è riferita all'introduzione di una cedolare secca sui redditi da affitto. Si tratta di un tema su cui richiamo l'attenzione dell'Aula, non fosse altro perché ciclicamente esso è un problema su cui trasversalmente tutti ci

vengono discusse e la condivisione si trova, ma il risultato non c'è mai. Quindi, vorrei che questa fosse la volta buona - per essere molto pragmatici - per riuscire a dare soluzione a questa problematica su cui sembrano esserci,

fuori dal reddito complessivo i redditi da locazione serva a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale su questa tipologia di redditi, perché si introduce un trattamento che è un trattamento fiscale oggettivo e non più soggettivo. questo sia sicuramente uno degli strumenti di decisa efficacia per contrastare il fenomeno delle locazioni illegali, che sappiamo esserci e che sappiamo essere ampiamente diffuso. Con questo strumento aiuteremo quindi ad accelerare l'emersione di quegli affitti che sfuggono al fisco e che - ripeto - interessano tutte le aree del nostro Paese. Peraltro, nel contesto macroeconomico ciò rappresenterebbe sicuramente anche un rilancio degli affitti a canoni ribassati in favore delle famiglie che più ne hanno bisogno, cioè quelle con basso reddito, che si trovano oggi a fare pesantemente i conti con un mercato immobiliare che, proprio per queste ragioni, dà decisamente poca concorrenza. Credo che i numeri

per cento delle famiglie in affitto ricade nella fascia di reddito sotto i 20.000 euro, e credo che esse sarebbero decisamente interessate agli effetti positivi che il nostro emendamento

delle differenze credo minimali, e su ci si può intendere. Possiamo proporre detrazioni fiscali per i locatori o delle deduzione fiscali? Su questo terreno ci si intende; l'importante è che si riesca su questo a un problema oggi paradossale: i redditi da locazione oggi hanno per i piccoli proprietari di appartamento costi fiscali ben superiori a quelli che hanno invece per

quando si garantiscono i saldi monetari, ma anzi nasce proprio garantendo i saldi monetari, e nasce perché di fronte al Paese e ai contribuenti ha la forza politica di spostare le risorse, e cioè di mettere in discussione gli 800 miliardi di euro di spesa pubblica per riallocarli in altre più efficaci ed efficienti funzioni. Questa è la politica economica: non la semplice salvaguardia (sacrosanta) dei saldi finanziari, non l'accettazione inerme degli andamenti tendenziali inerziali che ci provengono, purtroppo, dal ciclo economico internazionale europeo, ma la capacità e la volontà di incidere su quel 52 di prodotto interno lordo che rappresenta le decisioni collettive delle pubbliche amministrazioni e su quel 47 di prodotto interno lordo che rappresenta il totale delle entrate pubbliche, che chiamerei il totale delle uscite dalle tasche dei contribuenti, delle famiglie e delle imprese.

che individua due voci di spesa pubblica. La prima voce ha avuto una crescita anomala del cento negli ultimi cinque anni, e per due terzi si riferisce agli acquisti del settore della sanità, che non hanno nulla a che vedere con il Servizio sanitario e con la qualità della salute dei cittadini. I cittadini italiani credo che possano percepire che in questi anni quantità e qualità del servizio non sono aumentati del 50 per cento, come è aumentata la spesa.

in termini di uguale potere d'acquisto, considerando l'inflazione di questi anni, questo tipo di spesa pubblica, avremmo potenzialmente 20 miliardi di spesa in meno, senza toccare affatto la salute dei cittadini e i servizi sociali del settore di tutte le pubbliche amministrazioni. è quella dei cosiddetti fondi perduti. Nella contabilità pubblica italiana ufficiale ammontano a 44 miliardi di euro. Ogni anno,

Tali fondi perduti in questi decenni quanta produzione, quanta occupazione, quanti effetti sociali sul territorio, quanta chiusura del *gap* territoriale hanno prodotto? Ci sono varie stime che indicano valori molto prossimi allo zero. All'interno di questi 44 miliardi ci sono 15 miliardi che, tra conto corrente e conto capitale, vanno al servizio del trasporto pubblico locale. Vogliamo escluderli da qualunque intervento di contenimento? Bene. Ci sono 5 miliardi che sono i trasferimenti a sostegno delle ferrovie italiane. Vogliamo escluderli? Certamente è bene. Restano 24 miliardi di euro che vengono distribuiti a pioggia sotto forma di fondi perduti. Allora, la nostra proposta non è tagliare i sussidi, ma trasformare la forma con la quale la pubblica amministrazione sostiene la crescita, lo sviluppo e l'occupazione, cioè non fondi perduti *ex ante*, ma credito d'imposta, quindi sostegno alle imprese vere che stanno sul mercato anche dopo tre anni dall'aver ricevuto i soldi pubblici e non - come spesso accade - a quelle imprese che dopo tre anni,

l'indicazione politica, l'entità complessiva potenziale, allora queste risorse consentirebbero di dare un forte sostegno alle piccole e medie imprese,

un aiuto concreto alle forze di polizia e alle forze di sicurezza, per 2 miliardi di euro (un miliardo al Ministero della difesa e un miliardo al Ministero dell'interno, che compenserebbero i tagli effettuati); un miliardo alla ricerca per progetti congiunti università-imprese. L'aritmetica dice che la possibilità di intervenire su quel Moloch di 800 miliardi di spesa

Dopodiché ci rendiamo conto che forse un pizzico di prudenza circa la praticabilità immediata, soprattutto del contenimento della dirompente spesa per acquisto di beni e servizi (che spesso non rappresenta salute dei cittadini, ma salute di ben altre organizzazioni che sguazzano dentro quel tipo di spesa), potrebbe indurci a discutere le quantità. caso, non altrettanta prudenza è necessaria per la trasformazione dei fondi perduti in credito d'imposta, perché in quel caso l'effetto è automatico e aritmetico. Ogni trasformazione di fondo perduto in credito d'imposta, essendo il sussidio spalmato negli anni, determina evidentemente un risparmio di spesa. Questo è il quadro. Se vi fossero dubbi - e mi rivolgo al Governo e alla mia maggioranza - circa l'entità e la quantità,

per la semplice ragione che ciò che ho descritto è il programma elettorale, il programma di governo del centrodestra, del Popolo della Libertà, della Lega e del Governo Berlusconi.

Signora Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, i dati ufficiali dell'Agenzia del territorio, pubblicati nello scorso mese di luglio, indicano che in Italia 10.034.250 abitazioni che non risultano utilizzate dal proprietario, né affittate. Questa è l'entità (che appare per la prima volta) del parco potenziale degli affitti in nero. l'introduzione di una tassazione separata al 20 per cento per i piccoli proprietari e la deduzione di 5.000 euro l'anno per gli affittuari, con un onere al primo anno totalmente coperto senza un euro di deficit in più. Se dovessimo far prevalere la prudenza, potremmo partire con una riformulazione che al primo anno limiti a 1.000 euro la deduzione per gli affittuari. Non ci si venga a dire che è causa di ulteriore deficit pubblico, perché la verità è che se solo la metà degli affitti in nero emergesse dal secondo anno in poi, ci sarebbe un maggior gettito per l'erario di 2 miliardi di euro. È esattamente quello che è avvenuto negli anni passati

oltre a maggiore trasparenza e maggiore civiltà, con l'emersione di milioni di contratti di affitto.

Restiamo in attesa di una valutazione positiva almeno di questi emendamenti, che non comportano costi: occorre soltanto un pizzico di coraggio politico da parte

per contribuire ad arricchire il reddito della famiglia o le proprie disponibilità

L'unica considerazione che mi sento di fare, con l'emendamento 3.0.600 e con il successivo, è legata alla valutazione del diritto agli assegni familiari.

e al Governo di fare una valutazione attenta rispetto a questo vincolo. Faccio appello a tutti coloro che, nella maggioranza, hanno fatto riferimento alla famiglia affinché sostengano questo emendamento del Partito Democratico. *(Applausi

Mi riferisco a quei nuclei familiari che hanno nel loro interno un disabile gravissimo: parlo di un'invalidità al cento per cento, che sia tale da non consentire alla persona colpita dalla malattia nessuno degli atti normali della vita quotidiana.

a prescindere dall'età anagrafica, con il limite previsto di almeno cinque anni di versamento fatti in assistenza continuativa al grave disabile che si trova a casa. È evidente che questo emendamento ha un'utilità chiara chiara nei confronti di nuclei familiari già sfortunati e nella direzione di rendere più umana l'assistenza di un

questi ragazzi o ragazze disabili, nella maggior parte dei casi, vengono ricoverati in istituzioni sanitarie. E questo, in effetti, allo Stato costa molto di più di quanto si chiede con l'emendamento

Signora Presidente, onorevoli colleghi, gli investimenti in infrastrutture sono normalmente differenziati nel tempo: i progetti che oggi sono approvati vengono realizzati soltanto con molti

Nel merito, l'emendamento 3.0.7 si riferisce ad opere già previste in molte leggi dello Stato e che riguardano interventi infrastrutturali

sotto gli occhi di tutti la necessità di adeguare la rete delle Ferrovie dello Stato, soprattutto per quanto riguarda l'Alta velocità Milano-Verona e la realizzazione del terzo valico, ossia l'alta velocità Milano-Genova. quindi necessario ricapitalizzare la disponibilità di ANAS per poter realizzare la normale manutenzione per 1,2 miliardi di euro,

Baldassarri illustrando l'emendamento 3.0.10, che riguarda gli stanziamenti in favore della ricerca ed in favore delle forze dell'ordine e delle Forze armate. Per quanto riguarda specificamente il discorso degli investimenti in ricerca, credo che sia chiaro a tutti che ne va della competitività del nostro Paese. Nel 2009, nonostante la crisi, i principali Paesi occidentali

una accresciuta destinazione di risorse sia funzionale alla riforma dell'università, che arriverà tra l'altro proprio qui in Senato nei prossimi giorni, una riforma che fa fare un passo avanti molto importante e un salto di qualità al nostro sistema della formazione superiore, e che tuttavia necessita assolutamente di essere accompagnata da investimenti in istruzione superiore

affrontano il tema dell'IRAP e cioè il tema che ha dominato la discussione di politica economica in questo Paese nel corso degli ultimi mesi.

sotto il profilo economico. A questa domanda sia noi sia il centrodestra e il Governo diamo risposte sostanzialmente convergenti. In un contesto di ripresa incerta e debole ci aspettano sicuramente, soprattutto nei primi mesi del 2010, un forte aggravamento della disoccupazione e una ulteriore riduzione, indotta dalla disoccupazione crescente, della partecipazione alla forza di lavoro. In secondo luogo ci aspetta sicuramente, almeno per i primi sei mesi del 2010, il confermarsi di uno stato di *credit crunch*, cioè di sostanziale difficoltà delle imprese ad ottenere il credito sufficiente da parte delle banche per lo sviluppo della loro attività d'impresa.

che nel corso di questo 2009 hanno retto disperatamente, malgrado il fatturato fosse crollato e le condizioni per lo sviluppo della loro attività si fossero fatte molto precarie, in attesa di una ripresa che tarda, almeno per loro, così da convincere l'imprenditore piccolo e piccolissimo, che non ce la fa più, a dismettere la sua attività. A fronte di questa che ormai non è più una previsione, ma una certezza su ciò che accadrà nei prossimi mesi, diciamo che c'è bisogno di un sostegno alla domanda e all'infrastrutturazione materiale e immateriale del Paese che venga anche dagli investimenti della pubblica amministrazione, cioè dalla spesa in conto capitale. E abbiamo aggiunto che c'è anche bisogno di un sostegno all'attività d'impresa che - per quel che è possibile, nelle attuali condizioni di finanza pubblica molto difficili - riduca la pressione fiscale su tale E c'è bisogno - sempre per quel che è possibile nel difficile contesto di finanza pubblica - di un sostegno alla domanda dal lato dei consumi delle famiglie.

ha indicato un impegno preciso del Governo che dirige. Egli ha detto: in questo contesto mi rendo conto dell'urgenza di un intervento per la riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese.

signori del Governo, signora Presidente, come si diceva una volta quando si faceva qualche citazione latina, *hic Rhodus, hic salta*: adesso è il momento di verificare se queste sono parole vane,

oppure se, sia pure nel contesto di drammatica difficoltà nel quale si trova la finanza pubblica italiana, si ha la coerenza da parte vostra per fare un passo nella direzione giusta. Ho già avuto modo di notare che questa mattina la maggioranza e il Governo sono arrivati al punto di negare il loro consenso ad un emendamento che rifinanziava il fondo che è necessario rifinanziare per continuare nella detassazione della quota di salario da contrattazione di secondo livello che, colleghi di maggioranza, è l'unica (l'unica) iniziativa di riduzione della pressione fiscale che il Governo abbia assunto nel corso di quest'anno e mezzo

che aumentava le detrazioni e le deduzioni IRPEF a favore dei redditi medio‑bassi. Oggi pomeriggio arriviamo al tema dell'IRAP, sul quale vi presentiamo una proposta articolata su tre possibili interventi.

tra le assemblee degli artigiani e dei commercianti che rivendicano questa scelta nel Nord del Paese, ma anche nel Centro e nel Sud, esattamente allo stesso modo. proponiamo di eliminare dalla base imponibile dell'IRAP, che contiene l'intero costo del lavoro,

non avanziamo la proposta di eliminare dalla base imponibile dell'IRAP tutto il costo del lavoro per tutte le imprese, ma facciamo il primo passo: ci limitiamo ad eliminare la componente costo del lavoro dalla base imponibile dell'IRAP per le imprese di persone fisiche, non per le società di capitali. Certo, sarebbe meglio farlo per tutte le imprese perché, se è vero che siamo in una situazione per la quale temiamo un rinculo pesantissimo della crisi sul versante della disoccupazione, l'ideale sarebbe intervenire eliminando dall'IRAP il costo del lavoro nel suo complesso, ma sappiamo che questo non è possibile.

coperta con un aumento del deficit (non potremmo, perché l'emendamento sarebbe inammissibile); non copriamo con un aumento della pressione fiscale: copriamo con una riduzione della spesa corrente primaria, che è perfettamente praticabile e sostenibile a causa dell'onere limitato che questa proposta arreca. Potreste

signor Vice Ministro, la vostra legge sulla riforma della pubblica amministrazione, obbligandovi finalmente a dire che cosa vi aspettate in termini di riduzione della spesa corrente primaria da questo tipo di legge, dato che vi state rifiutando da un anno di associare a quella che chiamate la grande riforma della pubblica amministrazione un qualsiasi obiettivo di risparmio.

tutte le rappresentanze degli interessi economici dell'impresa di questo Paese, comprese le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, potranno piazzare i loro

Presidente Baldassarri, io voterò a favore del suo emendamento sull'IRAP e credo che il mio Gruppo farà altrettanto, intendiamoci bene, ma la nostra proposta, signori della maggioranza e del Governo, non potete respingerla in base all'argomento finanziario, perché nell'immediato non ha alcun costo. È una proposta che vi impegna a fare seriamente il mestiere che predicate di volere fare: cioè ridurre la pressione fiscale attraverso risorse reperite attraverso la riduzione della spesa corrente primaria. Se dite no, se il relatore dice no, se il Governo dice no non può usare l'argomento della insostenibilità finanziaria perché vuol dire che non riconosce nemmeno ciò che vi è scritto nell'emendamento. a voi non va bene nemmeno questo: ho presentato allora un altro emendamento che riduce l'IRAP, sempre dal lato della componente costo del lavoro nella sua base imponibile, attraverso il gettito di un'imposta nuova. Abbiamo tutti fatto dei comizi più o meno ascoltabili intorno all'orco feroce: i banchieri, i finanzieri. Il capo del banchieri, i finanzieri. Il capo del Governo inglese Gordon Brown ha recentemente presentato una proposta che che riguarda un'iniziativa a dimensione internazionale per un prelievo fiscale sulle operazioni finanziarie a breve. Molto più modestamente - non è un caso che io non sia il Capo del Governo inglese - ho avanzato un'ipotesi che riguarda la dimensione nazionale, che è la seguente: è vero o no, colleghi della maggioranza, signor Vice ministro, che nel corso della crisi abbiamo scoperto che lo Stato a spese dei contribuenti mette sulle banche, in

mettiamo una piccola imposta, che non è in realtà un'imposta, ma è un premio di assicurazione. Poiché noi, infatti, a spese dei contribuenti, abbiamo detto loro che non possono fallire, è come se avessimo garantito loro un'assicurazione. Per le assicurazioni di solito l'assicurato paga un premio.

il tema dell'IRAP è stato già affrontato ampiamente in Commissione ed è giusto anche in Aula fare un approfondimento. Anche la Lega Nord ha presentato una proposta in materia. È evidente a tutti che il problema di fondo è la copertura. Per non sapere né leggere né scrivere, abbiamo messo i fondi del FAS, ben consapevoli che tale copertura avrebbe trovato delle difficoltà, ma quanto meno esiste. Venendo al merito della questione, la nostra proposta - che poi è stata recepita per la parte propositiva, su cosa cioè si vorrebbe fare - contiene elementi che la differenziano un po' rispetto a quella del PD. il non determinare effetti sulle finanze regionali. Facciamo un ragionamento molto semplice, perché già si fece un errore sull'ICI , inizialmente dal Governo Prodi; poi - bisogna dirlo onestamente - si è proseguito su quella via, andando verso una sua eliminazione e non verso il meccanismo più corretto di mantenerla e consentire al contribuente di detrarla dal 740, per intenderci. Qual è il problema dell'IRAP? Faccio l'esempio della Regione Lombardia. La Regione Lombardia paga il 70 per cento della propria sanità proprio con l'IRAP. La stessa Regione partecipa al 53 per cento al Fondo nazionale di solidarietà per le Regioni che hanno difficoltà a coprire la spesa sanitaria. È evidente a tutti che sarebbe una follia dal punto di vista della Regione Lombardia eliminare *tout court* l'IRAP e poi, pur partecipando al 53 per cento al fondo di solidarietà nazionale, venire con il piattino a Roma a chiedere indietro i propri quattrini. Se si deve andare verso una modifica di tale imposta essa va fatta senza mettere in difficoltà e senza far saltare i conti

crea un altro problema, e questo è il primo punto. Il secondo punto riguarda l'entità. Sappiamo tutti che l'IRAP, definita in tempi non sospetti «imposta rapina», è una tassa molto odiosa.

è una battuta, però, tutto sommato, potrebbe anche funzionare. Venendo alla sostanza, come coprire questo abbiamo apprezzato l'apertura del vice ministro Vegas, che ha affermato che si può iniziare a ragionare su un'ipotesi di eliminazione per le aziende in perdita.

il punto è che siamo consapevoli che in tale fase non si può fare. Del resto, non muore nessuno, lo sappiamo che l'esame della legge finanziaria inizia a settembre e finisce a Natale; vedremo da qui a Natale che cosa succede. Vedo il collega Morando che sorride, però siamo veramente fiduciosi che, alla fine, qualcosa si riuscirà a fare. È chiaro che in questa sede sarà molto complicato: il problema è sempre e solo la copertura. Onestamente, a parte la copertura da noi proposta, quella

cento dell'inflazione programmata. È una proposta anche abbastanza forte, probabilmente se ne potrebbero fare anche di più forti, ma il senso è questo. Una volta per tutte dobbiamo cercare di affrontare il tema vero, il fatto cioè che oggi abbiamo un settore privato in estrema difficoltà. È il settore privato, infatti, che finanzia la spesa pubblica;

il disegno di legge sulla stabilizzazione dei precari e poi in futuro ancora di più, si renderà necessario ragionare seriamente sul comparto pubblico, perché se il settore privato soffre, alla fine mancheranno i quattrini per tenere in piedi la baracca.

La palla è nelle mani del Governo: vedremo quali saranno le modalità migliori per affrontare il tema vero, quello cioè di dare un po' di fiato alle nostre imprese. *(Applausi

in ogni caso, non c'è alcun dubbio che l'immissione nelle casse del sistema delle imprese di una liquidità di tale entità costituirebbe oggi una delle misure più efficaci per contrastare la crisi in atto e anche

si dovrebbe concludere che le cose non stanno così, nel senso che quello che noi proponiamo, cioè un'anticipazione e un'accelerazione di pagamenti di debiti già iscritti

il nostro emendamento, che prevede la cessione dei crediti alla Cassa depositi e prestiti, implicherebbe la sostituzione come creditore nei confronti delle pubbliche amministrazioni della Cassa depositi e prestiti alle imprese oggi creditrici. È giusta la posizione del Governo, ossia quella in base alla quale non è possibile provvedere a un massiccio pagamento, a una liquidazione immediata, per le ragioni che ho detto, perché si aumenta il debito? Analizziamo la situazione. La situazione è differenziata perché, ad esempio, per quanto riguarda il sistema degli enti locali, nei confronti dei quali vi sono crediti ingenti (in questa e in altre circostanze in quest'Aula abbiamo discusso diffusamente dei problemi legati al patto di stabilità), i ritardi nei pagamenti dei crediti vantati dalle imprese sono per larga parte originati dall'impossibilità

appunto, in molte occasioni di pagare le imprese per evitare di sforare il patto. In questo caso valgono tutte le considerazioni che abbiamo già svolto relativamente alla necessità e all'urgenza di mettere mano alla revisione del patto di stabilità interno, anche con misure tampone, in questa contingenza così difficile. Quindi, per quanto riguarda i crediti nei confronti dei Comuni, delle Province e delle altre autonomie locali, l'argomento è superabile solo mettendo mano al patto di stabilità interno. Naturalmente lo sforamento del patto di stabilità interno comporterebbe in via automatica anche l'accrescimento del volume globale del debito e, quindi, la posizione del Governo risulterebbe correttamente verificata. Analogo discorso vale nei confronti delle Regioni.

a ricorrere al meccanismo della cosiddetta cartolarizzazione, cioè alla cessione dei crediti alle banche, le quali diventano creditrici della Regione e pagano le imprese. In quel caso si è operata un'emersione dei debiti nei confronti del dei debiti nei confronti del sistema delle imprese per effetto, appunto, di questo meccanismo di cartolarizzazione. Si tratterebbe di verificare se esso ha dato frutti e se ha funzionato: a parte le gravi irregolarità e la *mala* *gestio* che si è verificata in qualche realtà territoriale, il meccanismo è corretto ed è analogo a quello che noi sostanzialmente proponiamo. Per quanto riguarda invece le amministrazioni centrali, signora Presidente, i noti SEC 95 della competenza economica ci dicono che è vero quanto segue: se il debito maturato, liquido, esigibile viene immediatamente pagato non c'è un effetto sull'indebitamento netto (perché, il criterio della competenza economica, oltre che di quella giuridica, implica già un avvenuto computo sull'indebitamento netto), ma c'è un effetto sul fabbisogno, sulla cassa e sul debito.

noi avremmo, con ogni probabilità, una crescita del debito pubblico di analogo o identico importo. È questa un'operazione sostenibile, sopportabile, opportuna, necessaria? Io ritengo di sì

prossimo o nel 2011. Quel debito che non si vorrebbe far emergere oggi per non peggiorare ulteriormente il già elevatissimo debito pubblico italiano comunque emergerebbe nei prossimi mesi e anni. Naturalmente, siccome i meccanismi viziosi - chiamiamoli così - si ripetono nel nostro Paese, è evidente che il non detto da parte della Ragioneria generale dello Stato

un volume di debito di eguale entità cosicché l'impatto sull'indebitamento sarà neutro nel senso che questo meccanismo vizioso si perpetuerà. paghiamo 30 si ricrea un volume di debito di 30 per debiti scaduti e non abbiamo un impatto immediato diretto aggiuntivo sul debito pubblico e sul fabbisogno, sulla cassa. È evidente quindi che la posizione del Governo, seppur fondata

permanentemente morose e di ritardi che permangono strutturalmente nelle amministrazioni pubbliche, nei pagamenti

alle pubbliche amministrazioni di certificare oggi l'ammontare dei crediti vantati delle imprese per lavori, forniture e servizi, alle imprese diamo la possibilità di cedere i loro crediti alla Cassa depositi e prestiti che dispone di un risparmio postale di liquidità

che è stato accantonato. Anch'esso contiene un argomento utilizzato più volte che riguarda la compensazione dei crediti delle imprese con i debiti tributari nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Dite qualcosa, assumete una posizione, facciamo qualcosa; se non lo fate, smettetela e smettiamola per favore (lo dico a molti colleghi, colleghi, soprattutto quelli della Lega Nord) di andare in giro per i territori riempiendosi la bocca del rispetto dei diritti delle imprese, dell'attenzione nei confronti del mondo delle piccole imprese. Se non facciamo questa operazione oggi, quando la facciamo? Ripeto, immettere una liquidità consistente oggi nel sistema produttivo italiano sarebbe la cosa meno onerosa e più efficace per contrastare la crisi.

È interesse dei titolari del contratto d'affitto ed è interesse anche dei proprietari delle case non regolarizzare la situazione.

Voi continuate a non rifletterci, noi continuiamo ad insistere; voi continuate a girare le spalle al Paese, ma tra un po' c'è qualcuno che vi rigira da quest'altra parte!

di grande soddisfazione né per la maggioranza né per l'opposizione, non ho alcun problema a svolgere una rapidissima premessa su argomenti che abbiamo già trattato ampiamente in Commissione e in parte anche in Aula. Lo faccio con disagio, perché non mi fa piacere dare la tagliola su una serie di emendamenti che sono condivisi dalla maggioranza e dall'opposizione e che però entrano in un ambito non di indefinitezza ma comunque quantomeno di incertezza sulle coperture. Immaginavo si potesse fare un maggiore sforzo

alcune caratteristiche generali degli emendamenti che sono stati sottoposti all'esame del Senato. In linea complessiva, gli emendamenti si possono dividere in due grosse categorie: nella prima si cerca di ridisegnare la manovra di politica economica, nell'altra si chiedono risorse per questo o quel settore secondo le le necessità dell'occasione. Circa il primo filone di emendamenti, invito l'Assemblea a considerare il fatto che la politica tenuta dall'attuale Governo - che certamente è poco

molti indicatori economici ci fanno notare come questa politica di estrema cautela e di rigore, nei limiti possibili offerti dal bilancio, evitando di nazionalizzare imprese o di entrare nel capitale del sistema bancario, ha consentito al Paese

allora riconoscere la positività di questo tipo di azione del Governo, che è stata proprio quella di non utilizzare la leva della spesa come hanno fatto altri Paesi i quali quando si uscirà dalla crisi si troveranno in condizioni ancora peggiori, perché dovranno far fronte ad un debito pubblico molto elevato e dovranno aumentare il ricorso al mercato o la tassazione, pregiudicando

Per quanto riguarda l'altro filone di emendamenti, quelli cioè che raccomandano di aumentare la spesa in questo o in quel settore, sono tutti complessivamente condivisibili, perché non

come in tutte le operazioni, soprattutto in quelle che si compiono in un contesto come la legge finanziaria, occorre ripartire tra i diversi obiettivi le possibilità finanziarie di cui si dispone, tenendo anche conto che

che valgano circa lo 0,5 per cento del PIL su base annua per poter recuperare gli ultimi anni, nei quali la crisi ha comportato scombussolamenti relativamente al debito e al *deficit*. Se manteniamo fissa la barra della politica economica del nostro Paese, possiamo realizzare la manovra che ci chiede l'Unione europea senza compiere manovre aggiuntive. Se invece aumentiamo la spesa in questo o quel settore,

per fare fronte alle maggiori richieste di spesa che andiamo accumulando. D'altronde, non si capirebbe perché lo Stato non si debba comportare come un qualunque individuo, che in momenti di difficoltà certo non aumenta la spesa e non va a chiedere soldi a prestito ma cerca di contenere le spese che

io personalmente - che l'IRAP è un'imposta sbagliata, perché anziché colpire i redditi, colpisce i costi; quindi è un'imposta che di per sé logicamente non regge mondo. Rimuovere questo tipo d'imposta, tuttavia, comporta un onere non irrilevante e quindi dobbiamo porci un problema di copertura che non può essere affrontato, come in molti emendamenti, con un semplice taglio lineare della tabella C, perché questa tabella è stata calibrata

Il problema principale, quindi, per la diminuzione della pressione fiscale - obiettivo al quale il Governo riconosce fondamentale rilievo e che è impegnato a perseguire nel corso della legislatura - se non ci vogliamo prendere in giro, è quello di trovare un corrispondente livello di spesa pubblica da tagliare effettivamente.

e anche il rinvio di spese al futuro forse è un metodo per navigare un po' meglio in queste acque agitate. Alcune questioni più limitate riguardano ad esempio il problema sollevato circa il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, certo un problema molto serio; però bisognerebbe tener presente anche il fatto che nella legge di assestamento per il 2009 sono stati disposti 18 miliardi aggiuntivi

all'erogazione di cassa abbiamo riscontrato un aumento che nel primo periodo si attestava intorno al 25 per cento di incremento rispetto al precedente periodo dell'anno scorso, e adesso è ulteriormente salito. Si tratta quindi di una misura che, pur necessitando

Per tutti questi motivi, riservandomi ovviamente di fornire risposte più precise quando esamineremo singolarmente gli emendamenti, credo che il complesso degli emendamenti che sono stati illustrati - certo molto interessanti per quanto riguarda le proiezioni e i desideri - si debba confrontare con la dura realtà della difficoltà della copertura finanziaria, e quindi forse non è questa la sede in cui essi possono essere approvati.

per far fronte ai problemi più urgenti, ad esempio quello dell'IRAP delle imprese in perdita; però dobbiamo tener conto che bisogna sempre affrontare i problemi con un approccio generale, perché certamente l'IRAP è un'imposta che molti hanno definito odiosa (non so se

bisogna stare attenti che sia equilibrata rispetto alla generalità dei contribuenti, altrimenti rischieremmo di creare scompensi che forse potrebbero essere non comprensibili.

i termini per la presentazione dei subemendamenti. Tuttavia, in queste agenzie di stampa, vedo un'indicazione esplicita secondo la quale questo emendamento conterrebbe norme che non sono state presentate né direttamente né indirettamente come proposte emendative in Commissione; quindi sarebbero completamente nuove. Le pongo quindi un problema che quest'Aula ha discusso nelle due precedenti legislature,

fa una verifica su questo punto per espungere le parti che non siano state presentate alla discussione precedentemente. Non dico esattamente identiche agli emendamenti presentati in Commissione, ma devono riguardare quei temi e quegli argomenti. Dal momento

naturalmente - come lei diceva - dovremo vedere il merito. Ne informerò anche il presidente Schifani; mi pare però, per quanto ci riguarda, che non sia neppure pensabile modificare regole che sono state assunte come comportamento nelle legislature precedenti.

noi ha un valore politico molto rilevante. Accanto alle tematiche concernenti il Mezzogiorno e il suo sviluppo e a quelle più squisitamente territoriali, il tema di una politica per la famiglia - cui il Governo ha fatto cenno molte volte, ma che attende di essere introdotto anche per consentire uno sviluppo della domanda, dei consumi - ci sembrerebbe una scelta opportuna. Mi perdonerete, quindi,

in realtà, stando stretti, si tratterebbe almeno di una decina. Allora, è chiaro che un emendamento di questo genere non avrebbe nessuna possibilità di successo per ovvi motivi di carattere finanziario.

Presidente, in questo caso la questione è un po' diversa, perché si tratterebbe di intervenire nel libero mercato e non credo che il Governo ne abbia l'assoluta facoltà, né ritengo che possa creare delle turbative di mercato. Sarebbe diverso fare un ragionamento nell'ambito della costituzione della Banca del Sud, di cui forse si potrà parlare presto.

una partita di banche, ma una struttura di credito che serva le famiglie e le imprese del Sud. Vorrei che questo fosse detto dal Governo in modo chiaro e solenne.

Presidente, l'emendamento 3.Tab.A.23 intende perseguire l'obiettivo assolutamente ragionevole di accantonare risorse per affrontare il tema del dissesto idrogeologico, sia dal punto di vista di una finalizzazione geografica che generale.

che riguarda la copertura finanziaria del sistema di protezione per i richiedenti asilo e per i rifugiati. L'attuale sistema di protezione nel nostro Paese per i richiedenti asilo e rifugiati ha una ricettività di circa 3.000 posti ed ha un costo annuale che si aggira intorno ai 32 milioni di euro.

che altrimenti il più delle volte scarichiamo sul sistema delle autonomie locali, che non hanno le disponibilità economiche e finanziarie per farlo e che quindi rischia di essere vulnerato. Poiché il Governo interpretato il sistema della protezione e della tutela dei rifugiati in modo "innovativo", utilizzando il sistema del trasbordo in Libia e quindi della garanzia in Libia, secondo il diritto libico, della protezione umanitaria,

che garantiscano il rispetto degli impegni internazionali da noi assunti. Questo è semplicemente il punto, Vice ministro; le chiedo dare una risposta su questo problema. Si tratta di impegni che abbiamo assunto solennemente in varie occasioni, l'ultima volta durante il Vertice de L'Aquila,

Signor Presidente, colleghe e colleghi, questo emendamento, che invito a considerare per una volta al di fuori dagli schemi maggioranza-opposizione,

senatore Vita,

Signor Presidente, in attesa che il relatore, la maggioranza e il Governo trovino un po' di soldi per le forze dell'ordine, noi chiediamo che almeno per il Fondo scorta del personale della Polizia di Stato si riescano a trovare 30 milioni di euro, che credo

intervengo molto brevemente per chiedere all'Aula di votare questo emendamento, teso a ripristinare il Fondo per le pari opportunità,

Non credo valga la pena di ricordare ai colleghi che da questo punto di vista l'Italia è purtroppo in un punto molto basso della graduatoria europea, piuttosto confutare quella che è stata una spiegazione: si dice infatti che non serve avere i fondi appostati alle pari opportunità a disposizione del Ministro per le pari opportunità e degli organi di parità, perché la politica di parità è trasversale. Questo è vero in teoria, però nella pratica sappiamo che tutta una serie di azioni vanno anche supportate con delle risorse. La politica di parità prevede di fare delle azioni positive a favore delle categorie (o dei generi, come in questo caso) discriminate, in sofferenza su alcune situazioni, in particolare nel lavoro. È inutile l'importante

cui non ci si può di occupare di queste cose e che quando sarà passata la crisi ci occuperemo di pari opportunità. Vale il discorso che abbiamo fatto sulla ricerca, l'università, l'innovazione e la banda larga: dipende anche da come usciremo come sistema Paese da questa crisi. Se puntiamo davvero sul grande capitale che abbiamo, mi riferisco al capitale umano, in termini di parità,

ulteriori 15 milioni di euro al ministro Bondi e quindi al nostro patrimonio culturale.

non ritualmente, ma perché in Commissione, quando ne discutemmo, si disse che per l'Aula, magari non per la cifra che qui è indicata, maggioranza e Governo condividevano con noi l'esigenza di un intervento a favore delle dotazioni finanziarie dell'ISTAT. Signor Presidente, si tratta di una questione tutt'altro che secondaria. La qualità della decisione politica, in materia di politica economica ma anche in materia di politiche sociali, dipende moltissimo dalla qualità delle informazioni circa la realtà del Paese di cui il decisore politico dispone.

loro fanno uno sforzo per migliorare la qualità delle informazioni che forniscono al Paese, quindi in primo luogo al Parlamento, ma sono in una situazione nella quale, lungi dal poter migliorare,

Ripeto, si potrebbe discutere della ricalibratura della cifra, però certo far passare anche questo momento senza un intervento di rafforzamento dell'ISTAT credo che sarebbe un'ennesima occasione persa per migliorare

gli altri sono stati falcidiati per motivi di preclusione da votazioni precedenti. L'emendamento in esame cerca di restaurare i fondi per gli alloggi e le residenze per studenti universitari, ma

ha rappresentato un attacco sostanziale, determinato e privo di ripensamenti all'importanza dell'istruzione, della trasmissione della cultura, della trasmissione della conoscenza e del peso fondamentale della ricerca nella nostra società. Siamo costretti a prendere atto che siamo di fronte ad una maggioranza e a un Governo che alimentano con una certa facilità una campagna di stampa che tende a presentare

caso non si tratta di essere ripetitivi sulla questione Abruzzo, anche perché è stato lo stesso Governo nazionale a sostenere che si tratta di una questione di rilevanza nazionale, nazionale, oppure di superare quella politica rigorista che punta alla necessità del controllo del debito o del deficit. Si tratta semplicemente di creare le condizioni per una pronta attivazione della ricostruzione pesante nel capoluogo di regione e nei comuni del cratere sismico attraverso un'operazione che anticipi

di intervenire nel corso del prossimo anno in tempi incisivi, ma ragionevolmente brevi,

delle grida d'allarme che provengono dal territorio. Non ultima, quella del Sindaco del capoluogo di Regione, che ha paventato il rischio di un grave dissesto finanziario del proprio Comune, anche alla luce di oltre 36 milioni di euro che mancano alle casse e alle disponibilità del Comune dell'Aquila. Signor Presidente, rivolgo pertanto un appello alla sensibilità dell'Aula. che - lo faccio senza alcuno spirito polemico - francamente non abbiamo compreso i criteri in base ai quali il relatore ha proposto l'accantonamento di alcuni emendamenti.

stati accantonati, nonostante le buone dichiarazioni del vice ministro Vegas: emendamenti presentati da componenti della maggioranza, che controribaltano totalmente la manovra finanziaria in atto, sono stati accantonati,

Con tali emendamenti intendiamo chiedere al Governo che le maggiori entrate derivanti dallo scudo fiscale siano prioritariamente dedicate al Fondo per l'occupazione.

che sarebbero seguiti interventi atti a compensare ed evitare condizioni di drammatizzazione, sul piano della ricaduta sociale, di quel tipo di iniziativa. Avendo mancato il Governo a quell'impegno,

per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato."».

Signor Presidente, è certo che la fase attuale della crisi è segnata drammaticamente dalla disoccupazione crescente, a cui si aggiunge la situazione davvero molto grave per tante famiglie conseguente ad anni di perdita di potere d'acquisto di salari e pensioni; una situazione che ha riflessi spesso drammatici sulla vita delle persone, come sappiamo bene, ma anche sull'economia generale, perché i consumi sono i due terzi del PIL: siamo ad un calo dei consumi *pro capite* di circa il 10 per cento, un dato rilevantissimo che è incredibile - ed io penso anche inaccettabile - non si cerchi di contenere e di contrastare con questa manovra finanziaria. Da questi elementi dovrebbe conseguire una priorità assoluta del tema lavoro e famiglia, con defiscalizzazioni per salari e pensioni, sostegno all'occupazione più debole ed a rischio e aiuti concreti alle famiglie per sostenere figli ed anziani. Questo emendamento, che noi ovviamente voteremo con convinzione, interviene certo anche parzialmente, ma con misure importanti in queste direzioni, prevedendo per prima cosa di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico che, come ricordavano altri interventi precedentemente, è ferma a più di 15 anni fa; di incrementare le detrazioni per i redditi fino a 55.000 euro, rispettando ovviamente i criteri di progressività come fissati delle norme, riconoscendo un credito di ammontare pari alla quota di detrazione per quei soggetti che sono fiscalmente incapienti; ancora, di aumentare la soglia degli importi deducibili per i mutui prima casa; infine, di prevedere forme di detrazione aggiuntiva per le donne lavoratrici per sostenerne ed incentivarne l'occupazione e aiutare così a conciliare la complessità dei diversi carichi di lavoro che pesano sulle donne. È una misura - ci tengo a sottolinearlo - che interessa circa 4 milioni di donne lavoratrici, in un momento in cui le difficoltà generali potrebbero pesare negativamente sulla tenuta di questo dato che anzi sarebbe interesse del Paese rafforzare ed ampliare. Ho sentito le dichiarazioni del relatore Saia, che in questo momento non vedo, imbarazzate e rassegnate nel dare il parere sugli emendamenti. Un po' lo capisco, anche se non condivido. Il vice ministro Vegas dice, in qualche modo gli entusiasmi sugli interventi sull'IRAP, che bisogna tenere conto anche delle esigenze dei redditi da lavoro e delle famiglie. Tutto vero; il risultato, però, piove su molti, e su qualcuno grandina, e non succede mai niente. Vorrei concludere il mio intervento richiamando un punto che è stato già ampiamente argomentato e non posso farlo ora in dettaglio: le nostre proposte hanno tutte profili di copertura seri ed affidabili. l'obiezione sulle scarse risorse non tiene: è un problema di priorità e di scelte, e quindi di una chiara responsabilità politica - se non sarà approvato questo emendamento - di questo Governo e della sua maggioranza.

Signor Presidente, credo che ci apprestiamo a chiudere velocemente questa legge finanziaria,

sull'IRAP avete annunciato prima un taglio di dimensioni consistenti che riguardava le piccole e medie imprese, poi siete passati ad un'ipotesi di detrazione delle perdite della base imponibile dell'IRAP, ad oggi non è pervenuto alcunché di concreto, se non l'ennesimo annuncio; infine, sulla famiglia le chiacchiere - come dicono da queste parti - stanno a zero. Non capisco quindi la ragione per la quale stiamo ancora qui qui a consumare questo rito: approvatevi la finanziaria; forse alla Camera qualcosa cambierà, ma il tema di fondo è che così non si va da nessuna parte, perché il Parlamento non ha più alcuna funzione ed alcun ruolo. Dico questo perché ritengo che obiettivamente

in esame, che non riguarda l'introduzione del quoziente familiare - perché è evidente che non c'è la copertura finanziaria per farlo, ed è uno strumento indispensabile che va introdotto progressivamente - ma prevede

con più figli, monoreddito e così via. Ora, non pretendo questo, perché è chiaro che il problema è tutto interno all'equilibrio della maggioranza e non riguarda la politica finanziaria ed economica di questo Paese; quindi, è tutta una partita che fra stasera e domani giocate all'interno della maggioranza, incrociandola con altre questioni che attengono al programma di Governo. Su temi centrali, però, che riguardano la famiglia italiana e sulla circostanza che in questo Paese un minore su sette vive al di sotto della soglia di povertà, non vi consentiamo

Accanto al mondo imprenditoriale ed economico e alla sofferenza che oggi presenta, accanto alle difficoltà del mondo del lavoro, l'altro grande tema che resta scoperto nel panorama italiano è quello della famiglia.

radicale e più efficace ma che comporta maggiori oneri dal punto di vista finanziario; si può scegliere un quoziente familiare parziale, oppure si può scegliere, ed è altrettanto efficace, una politica di sostegno dei redditi e dei servizi. Quindi ci sono diverse ipotesi. Peccato che la maggioranza,

la possibilità di svolgere un'attività lavorativa, vivono comunque una situazione di sofferenza e soprattutto di paura. Anche

in una richiesta di trasformazione in un ordine del giorno, per una ragione molto semplice: per come è definito, l'emendamento non contiene una prescrizione dettagliata delle misure di intervento sul carico fiscale delle famiglie, bensì

di vincolo politico e non certo alla non condivisione della proposta, credo che, com'è accaduto per uno degli emendamenti sulla materia che ho già trasformato in ordine del giorno, anche come segnale di disponibilità, piuttosto che incorrere in un'altra bocciatura di una previsione normativa che non avrebbe esito, sarebbe l'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno che ribadisca il valore politico di questo indirizzo, anche in linea con le richieste fatte dai colleghi dell'opposizione.

una predisposizione per l'accoglimento. Ma è inutile presentare tanti ordini del giorno sulla stessa

mentre gli altri Stati europei si sono ripresi. Per esempio, la Francia e i Paesi nordici, che tradizionalmente avevano meno bambini dell'Italia, hanno tassi di natalità più alti, perché hanno saputo gestire le politiche della famiglia.

e dare alle famiglie, e ai nostri lavoratori, la possibilità di sopravvivere e di vivere. Sappiamo benissimo che questa si basa anche sul lavoro delle donne,

tutto il sistema pensionistico, sanitario e di cura, tutto il sistema che si basa sul contratto di generazione. Ripeto, e non mi stancherò di farlo: sempre meno giovani dovranno sopportare il peso di una popolazione

al reddito familiare: mi sembrerebbe saggio. Per questo chiedo al relatore se è disposto a considerare un ordine del giorno in questo senso, che

i primi responsabili sono stati, invece, quelli dell'attuale Dicastero dell'economia. Perché, allora, per le entrate derivanti dai giochi questa equiparazione è andata bene, mentre non va bene per l'acquisizione del diritto all'erogazione degli assegni familiari, il cui limite di reddito è rimasto a 5 milioni delle vecchie lire,

a questo signor Governo, sono state alleggerite le tasche dei lavoratori a reddito fisso di un controvalore di 139 miliardi di euro, a vantaggio di coloro che adesso stanno facendo la fila nelle banche per il terzo riciclaggio di Stato, quelli cioè che riporteranno i soldi dai paradisi fiscali in Italia con

strumenti di sostegno al reddito delle famiglie sono già intervenuti, in fase di illustrazione, colleghi certamente più autorevoli di me. Io vorrei che si svolgesse un'ulteriore riflessione, perché, se è vero che sta sta trasparendo in queste ore e in questi giorni all'interno della maggioranza un certo strabismo politico tra quelli che sono gli annunci e i proclami e quelli che sono poi gli atti concreti che vengono messi in campo con questa manovra

non vorrei che i dati che si danno nei TG nazionali siano solo quelli che convengono al Governo. Nessuno di noi ignora che i dati EUROSTAT (che sono certamente più incrociati e più affidabili dei dati ISTAT) per quanto riguarda il rischio di povertà delle famiglie pongono in graduatoria l'Italia dopo la Lettonia, insieme alla Grecia e alla Spagna. Stiamo parlando di una manovra che non solo non dà qualcosa in più, cogliendo l'occasione di una crisi drammatica, ma destina quote in meno alle politiche per la famiglia. Vogliamo capire di quali entità stiamo parlando? Il Fondo nazionale per le politiche sociali

intervengo per sollecitare un incontro tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori della Fincantieri di Palermo, il Ministro dello sviluppo economico, unitamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e gli enti locali competenti. I lavoratori dei cantieri navali vogliono conoscere il loro futuro. Parliamo di maestranze di altissimo livello che danno lustro alla cantieristica navale dell'isola e all'intero Paese. È forte la preoccupazione per la possibilità di un processo di ristrutturazione del gruppo che possa modificare la cosiddetta *mission* produttiva sopprimendo le costruzioni navali e producendo il conseguente ridimensionamento degli organici. Vi è di più: in verità, la Fincantieri ha avviato finte trattative con promesse di commesse fantasma. La finiscano di raggirare gli operai con vane promesse e con carichi di lavoro inesistenti. L'unica scelta vera è arrivata: è la cassa integrazione, preludio della chiusura della struttura, alla faccia della crisi che sta finendo - dice taluno - o è psicologica, come afferma talaltro. In Sicilia quasi il 10 per cento delle imprese ha chiuso o sta chiudendo i battenti; parlo sia di grandi imprese che di quelle piccole sottocapitalizzate. Il cantiere navale di Palermo è componente storica dell'imprenditoria e dell'impegno dei lavoratori, alla stessa stregua degli operai della FIAT. Invito pertanto il Governo a non sottovalutare la vicenda la vicenda e a convocare nell'immediato le parti interessate.

Nel sollecitare la risposta del ministro Bondi, raccolgo anche il grido di allarme che proprio oggi ha rinnovato il sindaco di Arezzo, Giuseppe Fanfani, che paventa, a buona ragione, la perdita di un bene artistico e culturale del nostro Paese proprio alla vigilia delle celebrazioni vasariane. Mi sembrerebbe una cosa gravissima se dovesse accadere, e per questo sollecito una risposta urgente del ministro Bondi.

che ho l'onore di conoscere e che mi ha aiutato nella stesura della proposta di legge sul Garante dei detenuti, una lettera minatoria da parte delle Brigate rosse. Poiché egli

Questi sono atti negativi da non sottovalutare e da isolare. Ha fatto bene a portarli alla nostra attenzione. Il giudizio sulla concretezza è qualcosa che non ci riguarda: il fatto è grave che avvenga e deve essere stigmatizzato.